Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 ottobre. Rimane confermata per la seduta di oggi la discussione del disegno di legge in materia di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. Il calendario di questa settimana prevede, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, la discussione delle relazioni della Commissione antimafia sul riciclaggio e le infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito, la mozione Soliani ed altre connesse sul morbo di Alzheimer, la mozione Baio sulle etichettature dei prodotti alimentari per celiaci, nonché la mozione Marco Filippi sulla crisi del settore dell'autotrasporto. La prossima settimana, nell'intera giornata di martedì 11 ottobre, sarà esaminata, fino alla sua conclusione, la Nota di aggiornamento del Documento dì economia e finanza 2011. A partire da mercoledì 12 è prevista la discussione della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori e della Risoluzione della 14a Commissione permanente sulla Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, nonché la discussione della mozione D'Ambrosio Lettieri sull'acquisto dei farmaci via Internet. Il calendario dei lavori potrà essere integrato con informative del Governo relative alla vicenda Irisbus e ad altri settori industriali in crisi, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, nonché all'avvio dell'anno scolastico. Qualora la seduta di oggi pomeriggio non dovesse registrare i *quorum* richiesti, il Parlamento in seduta comune sarà nuovamente convocato domani mattina, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori. Pertanto, la seduta dell'Assemblea del Senato di domani comincerà alle ore 10.

la relazione proposta al disegno di legge e il breve testo del medesimo, composto da un articolo di un solo comma, potrebbero esaurire il ruolo del relatore. Mi corre, tuttavia, l'obbligo di rendere conto che la 13a Commissione permanente ha impegnato utilmente alcune sedute per una puntuale definizione del testo sottoposto oggi all'attenzione dell'Aula. Tra l'altro, la 13a Commissione ha tenuto conto di un ordine del giorno, approvato unanimemente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 18 novembre 2010, che - per facilità di consultazione - deposito agli atti, ma che ritengo utile in questa «La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, considerato che l'applicazione dei commi 5 e 12, dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativi alle forme di esercizio dell'attività venatoria in Regioni diverse da quella di residenza, ha originato differenti interpretazioni ed orientamenti, in rapporto alle previsioni degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; considerata la necessità di definire una lettura condivisa della normativa statale relativa all'esercizio del diritto di opzione delle forme di caccia nel territorio nazionale, al fine di coordinare le disposizioni della normativa nazionale di cui all'articolo 12, commi 5 e 12, della legge n. 157 del 1992, con le previsioni contenute nella disciplina legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; ritenuto a tal fine necessario proporre una norma a carattere interpretativo delle disposizioni nazionali sull'esercizio dell'attività venatoria al di fuori del territorio della Regione di residenza per chiarire il raccordo tra la legislazione nazionale e quella delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; chiede al Governo di promuovere l'adozione di una norma di carattere interpretativo delle disposizioni richiamate in premessa del seguente tenore: "Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso di consentire comunque l'opzione prevista dal comma 5 tra tutte le forme di caccia ivi indicate,

Per ulteriore e puntuale cognizione del contenuto del disegno di legge, che vuole appunto proporre unicamente l'interpretazione autentica di due commi della legge numero n. 157 del 1992 (i commi 5 e 12 dell'articolo 12), correlandone la comprensione ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della medesima legge, mi permetto di rinviarvi al testo dei medesimi. L'opportunità di una norma di interpretazione è in particolare riferibile ai numerosi procedimenti pendenti, conseguenti ad una innovativa interpretazione della normativa da parte degli addetti ai controlli in talune realtà provinciali nell'Appennino tosco-emiliano. Il disegno di legge aiuta a correttamente coordinare le precise disposizioni della legge n. 157 con le normative proprie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, pure esplicitamente richiamate dalla legge medesima. Questo disegno di legge non modifica in nulla la legge n. 157 sulla caccia, della quale la 13a Commissione sta da due anni ormai esaminando una ampia rivisitazione sulla base di numerosi disegni di legge già depositati, né intende modificare il riconoscimento delle potestà legislative riconosciute alle Autonomie speciali, quanto piuttosto sollecitarne la coordinata applicazione ai diversi casi che possono presentarsi concretamente. Sottolineo che la necessità di questa norma interpretativa, pur nella consapevolezza di quanto sia delicato e - come si dice - sensibile il tema, sollecita proprio una rivisitazione complessiva della legge n. 157, perché dopo quasi vent'anni occorre prendere atto anche dei numerosi cambiamenti intercorsi, sia in termini di sensibilità ambientale, di programmazione e di controllo, sia in termini di consapevolezza di ruolo da parte - mi pare - del pur difficile mondo Ma tutto questo richiede, appunto, ancora un approfondimento nell'ambito della 13a Commissione, e a questa prospettiva è sostanzialmente estraneo il modesto testo oggi sottoposto all'attenzione dell'Aula. Per esso desidero, infine, ringraziare la disponibilità del senatore Divina, primo firmatario dell'originario disegno di legge, che ha sostenuto i contenuti sostitutivi, nonché l'impegno del senatore D'Alì, presidente della Commissione, che ha costantemente operato in modo da rendere proficuo l'*iter* del disegno di legge.

Signora Presidente, colleghe, colleghi, credo che le motivazioni migliori per votare la richiesta di sospensiva siano proprio nelle parole che ha appena pronunciato il relatore.

e fino ad oggi non ha mai dato problemi interpretativi. Soltanto da pochi mesi, nel corso di quest'anno

del diritto del cacciatore, su domanda, di poter accedere ad altri ambiti. A chi non si intende di caccia forse dovremmo anche spiegare alcune cose: non è che i cacciatori possono andare in giro a sparare a qualsiasi cosa si muova. I comprensori o riserve di caccia che accettano cacciatori esterni sono riserve che hanno abbondanza di selvaggina e che devono fare prelievi sulla base di calendari venatori stabiliti non *ad libitum*, ma da organismi regionali dei quali fanno parte gli stessi organi di vigilanza regionale, le associazioni faunistiche e ambientaliste, esperti in materia di selvaggina e così via, che, studiando ambito per ambito e zona per zona, stabiliscono

punire persone che hanno rispettato la legge, che hanno fatto le domande previste, che hanno avuto le risposte e le autorizzazioni e che hanno pagato i permessi. Adesso, per una interpretazione confusa

ed inequivocabile - non possiamo penalizzare persone che in perfetta buona fede hanno fatto tutto ciò che la legge prescriveva. Spero che quest'Aula abbia minimamente capito di cosa si parla. Non c'entrano niente le obiezioni degli amici radicali, che possono rimanere della loro posizione anticaccia. Peraltro, non solo i contenuti sono sbagliati, ma anche la forma.

egregiamente. Mi stupisce, signora Presidente, che un'Aula del Parlamento, composta da più di 300 senatori, debba perdere il proprio tempo su una norma di buon senso, senso, che regolamenta una legge vecchia di 20 anni, praticamente nata ancora prima delle leggi europee. Stiamo cercando di normalizzare dei contenziosi che si stanno perpetuando da anni su tutte le Regioni, e non solo in Trentino.

devono continuare a lottare anche in queste Aule del Parlamento, quando i cittadini italiani con

e convintamente voterò contro la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. credo infatti che oggi vada almeno difesa l'integrità,

credo infatti che oggi vada almeno difesa l'integrità, più volte aggredita e messa in discussione, proprio della legge n. n. 157 del 1992, in cui si definisce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse nazionale ed internazionale. norma, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza della conservazione della fauna selvatica. Già nel 1992 si attribuì alle Regioni il compito primario di emanare norme relative alla gestione e alla tutela in conformità delle leggi e delle convenzioni internazionali. Le Regioni tutte, dunque, hanno compiti precisi che non possono ancora una volta esser aggirati. È anacronistico, oltre che assai grave, che proprio questo Governo, sedicente federalista, tradisca ancora una volta le autonomie territoriali

la senatrice Poretti diceva che i modi potevano essere diversi: si poteva attivare una sanatoria, si potevano mettere le mani nelle tasche proprie (sappiamo che di norma questo Governo le mette nelle tasche altrui, ma nel caso specifico

potrebbero - e potranno - così legittimamente eludere l'obbligo prioritario di conservazione del patrimonio faunistico che spetta all'autorità statale, cui è affidato il compito, secondo la Corte, di adottare i criteri minimi di tutela ai fini alla conservazione, realizzandosi così un'evidente disparità tra le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. Pertanto, il ricorso alla legge di interpretazione autentica per dare un'interpretazione difforme dalla legge in oggetto è è un atto abnorme e incostituzionale in quanto le norme interpretative non possono violare i limiti generali che attengono alla salvaguardia ambientale, oltre che ai principi costituzionali. Resto convinta che una norma interpretativa, per essere costituzionalmente legittima, possa essere adottata dal legislatore solo quando sussistano incertezze sulla sua applicazione o contrasti giurisprudenziali, tutti presupposti assolutamente mancanti nel caso in questione, dove la legge n. 157 del 1992 disciplina in maniera univoca l'attività venatoria, sia per le Regioni a Statuto ordinario che per le Regioni a Statuto speciale. Il 2422 risulta essere pertanto, oltre che incostituzionale per i profili citati, uno strumento surrettizio per aggirare le procedure ordinarie di approvazione delle leggi. Si tratta in tutta evidenza di un attacco al cuore della legge n. 157 del 1992, con il chiaro intento di allungare i tempi di caccia. Si tratta di una forzatura culturale e politica che manomette l'unica legge italiana di tutela della fauna selvatica, che causerà senz'altro, come già detto, un vero e proprio caos in tutte le Regioni, dalle quali non è improprio pensare che si susseguiranno ricorsi, pressioni e contenzioni senza fine.

un regalo rispetto a numerosi e reiterati comportamenti scorretti che li hanno visti protagonisti nell'ultimo periodo, e alle conseguenti sanzioni, che questi dovrebbero pagare, anziché farsi fare leggi apposite per non rispondere alle giuste punizioni.

riflettere. A questo punto entriamo anche nel merito, perché il metodo credo che comunque occorra sottolinearlo. L'avevamo sottolineato nella questione sospensiva ricordando gli articoli del Regolamento del Senato

che cerca di interpretare una legge, ed alla fine parla testualmente di un'interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge sulla caccia.

più felici. La legge n. 157 del 1992 parla chiaro e stabilisce il principio dell'opzione esclusiva di caccia, vale a dire la possibilità per chi spara di esercitare una sola delle forme di attività venatorie previste: vagante in zona Alpi, da appostamento fisso o nell'insieme delle altre forme consentite. I cacciatori trentini in questione erano stati multati perché avevano esercitato la caccia in altre regioni, pur avendo scelto quella in zona Alpi. Se questo principio non ci va bene, lo si cambi

è - si potrebbe dire con un'interpretazione autentica - un'ingiustizia anche nei confronti di chi, svolgendo un'attività venatoria, osserva la legge.

perché si consente di violare una legge, di andare contro una legge perché c'è qualcuno, qualche santo in Paradiso, che probabilmente non è san Francesco, se mai esiste un Paradiso, che poi protegge la sospensiva non andava bene; la senatrice Amati vi ha illustrato anche una serie di dubbi di costituzionalità (e avevamo anche pronta una pregiudiziale di costituzionalità),

hanno votato contro la sospensiva, perché, in qualche modo, ci ripensino ed entrino davvero, non nel merito del tema "caccia sì"-"caccia no", ma nel merito di come si fanno le leggi e di come le istituzioni debbano essere utilizzate, *in primis* da noi.

la pregherei, cara senatrice, di non permettersi più, in queste Aule del Parlamento, di portare offesa ai cittadini cacciatori che, con le tasse che pagano, contribuiscono a pagare anche il suo stipendio.

mi dispiace che il dibattito si radicalizzi su queste posizioni. Sembra qui di doversi schierare a favore o contro la caccia.

la popolazione di daini, di caprioli e soprattutto di cinghiali è esplosa. Pertanto quelle riserve, traboccanti di selvaggina, avevano estremo piacere di poter invitare i cacciatori, altrimenti avrebbero dovuto prevedere piani di abbattimento straordinari.

l'organo gestore di una certa riserva della regione appenninica autorizzava il cacciatore all'uscita per quella giornata,

il danno oggettivo, finanziario ed economico) su persone incolpevoli. Quest'Assemblea è chiamata a dire se è giusto che persone incolpevoli debbano essere punite, come, se noi non facessimo niente, sarebbero inevitabilmente punite. in certi ambiti si sono bloccati i provvedimenti, dilazionati i tempi, sapendo che su questa norma probabilmente si sarebbero trovate una formula, una via d'uscita. Addirittura, le prefetture tengono fermi i provvedimenti sanzionatori sanzionatori e amministrativi in base ai quali se uno viene condannato ci sarebbe una pena accessoria, probabilmente anche la sospensione del porto d'armi e del permesso di caccia per un certo periodo. A cascata, poi, il disastro farebbe a sua volta ancora più danni. a questo punto: abbiamo capito che c'è un sistema normativo vulnerabile, con pecche e falle. Noi in questo momento non abbiamo il tempo di riprendere in mano tutta la legge; prendiamo allora in mano l'aspetto normativo e sanzionatorio, diamo una risposta, decidiamo se è giusto darla, a chi incolpevolmente si è trovato sotto un fuoco di fila perché per vent'anni ha fatto sempre una cosa che la legge gli consentiva e per vent'anni la cosa è andata sempre regolarmente, mentre l'ultimo anno qualcuno ha dato letture diverse della stessa norma e dei

l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 rappresenta uno dei capisaldi della legislazione venatoria italiana, allorché, prevedendo le opzioni di caccia, rafforza il principio del rapporto cacciatore-territorio quale aspetto fondamentale per una buona gestione del territorio e una adeguata tutela della fauna. Al tempo stesso riconosce giustamente una specificità a particolari tipologie di caccia quali sono quelle da appostamento fisso, quelle che si esercitano in zona Alpi e per risulta le altre forme di caccia. La modifica di questo articolo avrebbe richiesto una discussione molto più larga ed approfondita perché si tratta di aspetti di ordine generale che riguardano l'intera normativa. Qui si ricorre alla modifica dell'articolo 12 per risolvere - come sottolineato più volte dai colleghi che mi hanno preceduto - il problema che hanno avuto un centinaio di cacciatori multati perché trovati ad esercitare la caccia fuori dalla propria regione di residenza in violazione violazione dell'opzione di caccia prescelta - quella della zona Alpi -anche se autorizzati dalla Regione ospitante. Credo che ben altre soluzioni potevano essere trovate. In questo modo, non solo si estende a tutte le Regioni a statuto speciale una deroga, che peraltro non tutte hanno richiesto; non solo si intacca il principio basilare della caccia sostenibile e popolare del nostro Paese, attivando meccanismi consumistici che hanno a che vedere con l'esigenza di conservazione della fauna; non solo si sceglie una strada unilaterale che presuppone la legalizzazione di un privilegio solo per una piccolissima fetta di cacciatori a discapito della stragrande maggioranza, ma si forza la legislazione in una logica di deregolamentazione che più volte, anche in questa sede, per iniziativa del Gruppo del Partito Democratico abbiamo attentamente e fermamente evitato. Noi siamo dalla parte di una caccia rispettosa degli equilibri naturali, delle indicazioni della scienza e delle prescrizioni comunitarie e, in questo senso, abbiamo combattuto gli opposti estremismi utili solo a fomentare lacerazione sociale e ad accrescere un conflitto di cui il Paese non ha davvero bisogno. Alcune esperienze virtuose sui territori dimostrano - e qui parlo anche per diretta cognizione di causa e per esperienza personale personale condotta in passato in un pezzo di territorio del Mezzogiorno - che è possibile trovare un giusto equilibrio che tenga debitamente conto, coniugandole tra loro, delle diverse esigenze: quelle dell'associazionismo ambientalista, quelle dell'agricoltura e quelle del mondo venatorio. Sulla vicenda che è a monte del provvedimento che ci occupa non ci saremmo sottratti se fossero state affacciate soluzioni diverse, direttamente collegate alla sanatoria di un contenzioso amministrativo. Ma la linea che oggi la maggioranza sostiene ci fa arretrare sul piano sociale e anche - se mi è consentito - sul piano culturale e, per risolvere una questione vera,

Signora Presidente, non so se il senatore Carrara è ancora in Aula, visto che lamentava la perdita di tempo e magari non lo vuole perdere davvero. Noi, in effetti - concordo con lui - stiamo perdendo del tempo perché si

il suo atteggiamento benevolo nei confronti delle questioni da sanare, bastava fare una sanatoria (contro la quale noi ci saremmo comunque schierati), mettere da parte gli interessi di un centinaio di persone

le istituzioni ad essere offese da questo uso *ad categoriam* che viene continuamente fatto. Questo si faceva anche negli anni '20 e '30, ma non è andata troppo bene all'epoca.

cioè un'avversione, legittima, nei confronti dell'attività venatoria. Quello che mi dispiace - mi rivolgo al collega Andria - che chi evoca una equidistanza tra gli opposti estremismi non abbia voluto approfondire il testo di cui parliamo, le ragioni per le quali il disegno di legge è di interpretazione autentica, la storia di questi 19 anni di applicazione degli articoli 12 e 16 della la totale disparità di comportamento delle Province italiane circa l'interpretazione di questa norma ma di questo, ahimè, nessuno ha voluto prendere visione - l'appello all'unanimità delle posizioni di Conferenza Stato-Regioni, Governo e Parlamento al fine di fornire un'interpretazione autentica della legge.

che avesse fatto richiesta ad un ambito territoriale di una Regione diversa dalla sua e che fosse stato accolto, venisse multato. Non è mai capitato.

sulla base di un'interpretazione innovativa dell'articolo 12 della legge n. 157 che mai, prima dell'anno scorso, è stata data in Italia. E voi davvero pensate che i cacciatori trentini vadano fuori regione soltanto in quattro province?

e abitualmente faccio tre-quattro giornate di caccia in Toscana, un paio in Veneto e una in Sicilia. Nessuno si è mai sognato di multare il sottoscritto o gli altri cacciatori per un semplice fatto,

cacciatore trentino, invece di richiedere il tesserino toscano, si è presentato con il tesserino del Trentino ed è stato multato in due province su sette.

questa eccezione, che ha riguardato solo 100 persone e solo in quattro province, alla regola di un'applicazione di una legge che per 19 anni è stata la stessa e che continua ad essere la stessa per tutto il territorio nazionale e per tutti i cacciatori provenienti da qualunque provincia d'Italia. E, se non fosse così, non ci sarebbe stato dai rappresentanti di quelle due Regioni, Toscana ed Emilia-Romagna, il voto favorevole all'unanimità in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla richiesta al Parlamento di interpretazione autentica. allora di che cosa stiamo parlando e che scenari stiamo evocando rispetto alla violazione di autonomia, alla violazione della territorialità del cacciatore e alla violazione dell'applicazione della legge, se rispondiamo all'appello fatto dalla Conferenza Stato-Regioni che incita il Parlamento italiano a

del provvedimento che ci accingiamo a votare oggi, cari colleghi, e mi stupisce ancora una volta su questo tema anche la totale disarticolazione dal sistema degli enti territoriali, dalle Regioni, dalle esigenze del territorio di una parte del Parlamento che fa finta di non vedere che tutte le Regioni italiane, comprese quelle governate dal proprio partito, hanno chiesto al Parlamento un intervento per un'interpretazione autentica.

le forze dell'ordine, il Corpo forestale dello Stato, le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile dell'ENPA, le guardie delle associazioni ambientaliste, le guardie delle associazioni venatorie e la Polizia provinciale. In questo contesto complessivo di 11 soggetti che fanno vigilanza, si è creata una crepa nel sistema, con un'interpretazione che è capziosa, e per questo interveniamo. Interveniamo, in sostanza, contro un'interpretazione capziosa che dopo 19 anni scopre che vi sarebbe un vincolo che la legge non dice e che dopo 19 anni individuerebbe soltanto in quattro province un divieto che nel resto d'Italia non c'è. Ebbene, riportato a questo tema, e solo a questo tema, e richiamato - credo - alla responsabilità di tutti che vi è un documento della Conferenza

che, proprio nel caso specifico, ha i requisiti dell'interpretazione autentica, proprio perché vi è disparità di trattamento e di interpretazione e proprio per il fatto che in quattro province un organismo di vigilanza pretende di sanzionare ciò che, nelle medesime province, gli altri organismi di vigilanza non sanzionano e che nel resto d'Italia nessuno si è mai sognato di sanzionare. Ritornando a questo provvedimento, che è davvero piccola e poca cosa, credo che potremo ciascuno con tutte le sue ragioni - riservare ad altri scenari e ad altri provvedimenti l'appassionante dibattito su «caccia sì-caccia no» e oggi fare il nostro mestiere di legislatori, che talvolta è anche quello di corrispondere ad una richiesta di interpretazione che arriva dalle Regioni italiane per dare una uniformità di comportamento e di interpretazione ed evitare il caos delle piccole Repubbliche o

i cacciatori multati nelle quattro province avevano fatto richiesta all'amministrazione provinciale dell'accesso al territorio di quelle province. L'articolo 14 dice che, fuori dalla propria regione, uno deve domandare, e gli si può rispondere di no, perché il governo dell'attività venatoria di ogni singola provincia consente di contingentare il numero dei cacciatori provenienti dall'esterno. Questa è la legge n. 157, così come si applica. E il paradosso dei paradossi è che queste persone ammesse all'attività venatoria dall'amministrazione provinciale sono multate. sono multate. Ne va anche della credibilità di questo ente che, a istanza e dietro pagamento di una tassa di concessione, ha consentito loro l'accesso. Ma di che cosa stiamo parlando, collega Poretti?

il dibattito su questa questione alla piccola cosa che è, perché è tale; piccola cosa dietro la quale, tanti o pochi che siano, del Trentino o della Sicilia, c'è un gruppo di cittadini che è stato trattato in maniera diversa dal modo con il quale sono stati trattati tutti gli altri cittadini italiani, e ci sono - lo ripeto fino alla nausea - le Regioni italiane che ci chiedono di chiarire l'applicazione della legge. Se volessimo tornare in questo alveo, forse oggi il Parlamento farebbe un servizio utile al Paese.

Signora Presidente, senatrice Amati, dove è scritto che le norme delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome siano meno ferree nella tutela del patrimonio faunistico?

«La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente». E poi: «La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale». In realtà, la norma di interpretazione autentica contenuta in questo disegno di legge è necessaria solo per favorire la connessione fra gli articoli 12 e 14 della legge n. 157, che parlano proprio delle competenze dei diversi livelli. Senatrice Poretti (se mi è permessa una digressione): San Francesco è patrono d'Italia, non degli animali. «L'Osservatore Romano» di oggi ci aiuta molto in questa lettura. Mi piace far echeggiare in questa sede il nome di monsignor Giuseppe Placido Nicolini, di Trento, che fu vescovo di Assisi per mezzo secolo, tra l'altro con grandi riconoscimenti, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Fu il vescovo Nicolini a proporre a Papa Pio XI l'atto, che fu poi tra i primi di Papa Pio XII nel 1939, di proclamare San Francesco patrono d'Italia. Se poi tutte le riflessioni che ho provato a fare hanno un senso, mi sembra riduttivo definire questo certamente faticoso e per certi versi inopinato impegno del Senato su questo piccolo disegno di legge come l'impegno su una leggina per quattro cacciatori per fare loro un favore. Quantomeno vorrei restasse agli atti che io cacciatore non sono. Il senatore Carrara ha voluto ricordarci che si tratta di una norma di buon senso. Al senatore Divina vorrei riconoscere il merito di aver accettato una rivisitazione importante del suo originario disegno di legge: quello sì toccava la legge n. 157, modificandola. Il senatore Andria proponeva soluzioni diverse, come un'eventuale sanatoria, ma proprio qui si propone un'interpretazione autentica per lasciare intatti i principi e le questioni affrontate positivamente dalla legge n. Sotto questo profilo, il senatore Orsi ha spiegato ordinatamente le motivazioni prossime di questo provvedimento, segnalando l'eccesso delle interpretazioni ultimamente intervenute sul territorio.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri : - sull'emendamento 1.2 parere contrario, in quanto l'effetto che si produrrebbe è suscettibile di differenziare, in modo irragionevole, le forme e le condizioni di autonomia che la Costituzione riconosce, nella medesima intensità, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; sull'emendamento 1.101 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista appare ultronea o, in caso contrario, potrebbe essere suscettibile di una interpretazione lesiva delle competenze regionali in materia; - sui restanti emendamenti parere non ostativo». «La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.0.100, parere non ostativo, a condizione che sia inserita una clausola che espliciti la necessità del consenso della Regione interessata in materia di accesso dei cacciatori in tutti gli ambiti territoriali costituiti per l'esercizio dell'attività venatoria; sull'emendamento 1.0.101, parere contrario, in quanto le norme ivi contenute prevedono, a carico delle Regioni, obblighi che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni stesse, devono essere configurati come mere facoltà;

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione che sulla proposta 1.0.101, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2». vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola secondaria statale di I grado «Carmine Sylos» di Bitonto, in provincia di Bari, ai quali diamo il benvenuto.

non parliamo del sangue degli animali, ma di quello degli uomini e delle donne. Quest'anno le vittime

un colpo dal fucile: ferito alle gambe l'amico a Sassoferrato». «Ragusa - Cacciatore modicano colpito dalla scarica di piombo di un parente in un incidente di caccia». «Como - Padre impallina la figlia cacciatrice, incidente di caccia a Lierna». «Varese - Incidente di caccia, trentenne rischia di perdere un occhio». «Piacenza - Fossadello: impallinata alla gamba mentre corre la gara, indagano i Carabinieri». «Viterbo - Montalto di Castro. Lo scambia per una quaglia e gli spara». «Milano - Monza Brianza: Spara alla lepre e ferisce un cacciatore. L'uomo raggiunto dal colpo rischia di perdere la vista». «Arezzo - Muore cacciatore di 54 anni colpito da una fucilata». Non sono parole mie: sono i titoli dei giornali locali che hanno riportato i danni collaterali della caccia.

pur riferendomi alla richiesta della 1a Commissione della clausola aggiuntiva e pur avendo esso un'attinenza con l'impianto del disegno di legge oggi in discussione,

per ragioni tecniche di merito che spiegheremo tra breve e per ragioni più generali connesse alla necessità di un quadro normativo certo, stabile ed applicabile, in una materia sulla quale l'Italia ha da tempo un pesante contenzioso con le istituzioni comunitarie.

e comunque con modalità non in contrasto con i superiori valori di cui all'articolo 9 della Costituzione. Ogni strappo procedurale inferto al già problematico equilibrio della disciplina vigente vedrebbe sempre la netta contrarietà del nostro Gruppo. Il disegno di legge sul quale ci si accinge a votare era volto, almeno nella sua formulazione originaria, a modificare direttamente la legge n. 157 del 1992 per esplicitare il diritto a cacciare in ambiti diversi da quello di appartenenza del richiedente, previa autorizzazione degli organi di gestione della riserva o di ambito. Tale proposta era nata dal fatto che nell'ultimo anno sarebbero stati rilasciati verbali sanzionatori di autorità di controllo venatorio nei confronti di cacciatori provenienti dalla «zona Alpi», i quali esercitavano l'attività venatoria in zone diverse dalle Alpi. L'intervento normativo iniziale avrebbe avuto l'effetto di eliminare radicalmente il criterio dell'esclusività della scelta di una delle diverse forme di caccia elencate all'articolo 12, comma 5, della legge ed avrebbe fortemente, se non inesorabilmente, indebolito lo spirito della tutela, finendo peraltro con l'applicarsi ben oltre la zona alpina. La Commissione ha invece proposto all'Assemblea una interpretazione autentica del principio di esclusività, facendo riferimento ai poteri normativi riconosciuti alle Regioni a statuto speciale. L'Italia dei Valori, anche comprendendo le difficoltà applicative registrate, non conviene con tale soluzione, pur rilevandone la minor invasività rispetto alla prima stesura. Il nostro ragionamento ha una valenza anzitutto giuridica.

al fine di contenere la soggettività dell'interprete e rendere il più possibile oggettivi e prevedibili i risultati dell'interpretazione, ha disciplinato l'attività interpretativa nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, indicando espressamente i criteri cui il giudice deve attenersi. Il sistema giuridico ha quindi già previsto, oltre alle sedi applicative proprie (vale a dire l'attività giurisdizionale e quella amministrativa), anche i criteri interpretativi di norme che dovessero risultare poco chiare. Noi non possiamo auspicare una continua rincorsa del legislatore a modificare o interpretare le leggi a seconda dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in un dato momento (che peraltro concerne solo le parti in giudizio e non la generalità dei cittadini) o, come nel nostro caso, in base ad atti meramente amministrativi posti in essere in una singola parte del territorio nazionale, poiché la legge già contempla le sedi cui rivolgersi ed i modi per impugnare le sanzioni ritenute illegittime. Ciò detto, quando il legislatore ricorre ad una interpretazione autentica non dovrebbe mai incorrere nel medesimo difetto di opacità della norma che intende interpretare. A tale proposito, la disposizione in esame presenta un difetto di base: essa interpreta la legge vigente in riferimento alla normativa delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale (quasi che l'arco alpino fosse solo a queste ultime delimitato). Da un lato, emerge un contrasto tra la legge dello Stato e le norme degli Statuti speciali, con necessario corollario di conflitto suscettibile di essere portato di fronte alla Corte costituzionale; dall'altro, non si consegue neppure l'allineamento della disciplina sanzionatoria fra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale. Il rischio è quello di introdurre nell'ordinamento una chiave innovativa che la Corte costituzionale potrebbe non ammettere. Per costante giurisprudenza costituzionale va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di modo che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella interpretata e l'altra interpretativa che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. Una interpretazione innovativa sarebbe illegittima. La norma interpretativa, inoltre, assume per sua natura valore retroattivo in deroga al generale principio di cui all'articolo 11 delle preleggi. Dovrebbero perciò essere valutati, in assenza di dati, anche i riflessi della nuova legge sui procedimenti futuri ed in corso. Il rischio principale, a nostro modo di vedere, è che la norma finisca comunque con l'indebolire l'esclusività della forma di esercizio della caccia stabilita dalla legge e che, perciò, essa non sia utile neppure a chi esercita l'attività venatoria. L'occasione odierna è utile anche per ricordare che interventi normativi estemporanei che inseguono singole controversie, quasi mai riescono a risolvere i problemi concreti. In materia di caccia ciò è avvenuto anche con la recentissima sanzione avente ad oggetto l'abbattimento di esemplari di animali. Sul nuovo articolo 727-*bis* del codice penale si è già pronunciata criticamente la dottrina e sarà probabilmente necessario correggerlo per ovviare al mancato coordinamento tra questa disposizione e la normativa previgente, che rischia di rendere peggiorativa la legge da poco in vigore. In conclusione, rileviamo che un intervento legislativo animato dall'intento di dare soluzione legislativa a problematiche che già dispongono di una sede amministrativa o giurisdizionale idonea per essere affrontate e risolte non risponde ad una particolare urgenza. Preso atto che molto più grave sarebbe stato ogni tentativo di deregolamentare aspetti sostanziali della disciplina venatoria in modo da svuotarla di fatto, ribadiamo quindi una valutazione contraria sull'utilità del provvedimento in esame, stante il carattere residuale che il ricorso all'interpretazione autentica dovrebbe sempre avere, nonché della necessità di ponderarla più ragionevolmente di quanto non si sia potuto fare in questa occasione.

questione, che è stata giudicata a livello di Conferenza un problema cui dare risposta, perché troppo era il caos. Ribadisco fino alla nausea che quelle persone che oggi sono state multate - e per le quali vedremo di trovare una soluzione - hanno esercitato un diritto *ex lege*; nulla hanno violato della legge se non che per diciannove anni questa è stata interpretata in una certa maniera su tutto il territorio e adesso, soltanto in due province d'Italia

difficoltà a pagare queste sanzioni. Ribadisco che non parliamo di provvedimenti ideologici: la caccia non è di centro, di destra o di sinistra, ma, se me lo consentite, essa è stata una grande livella sociale, è stata una grande livella sociale, se pensiamo che fino a non poco tempo fa era appannaggio soltanto della nobiltà, che si esercitava in riserve private. La gestione della fauna pubblica, a seguito delle leggi dello Stato e delle Regioni che hanno consentito venatorio è stata pertanto una grandissima operazione sociale. Una seconda azione sociale la fanno i cacciatori che, con diritto e autorizzati,

gestiti anche con organi ai quali partecipano movimenti ambientalisti, danno pertanto la massima garanzia dell'equilibrio venatorio. I cacciatori che vanno a fare queste operazioni, del resto, portano anche denaro, da utilizzare per operazioni di ripopolamento

Signor Presidente, colleghi, credo che, a seconda che lo leggiamo con maggiore o minore malizia, questo disegno di legge rappresenti un caso tipico di eterogenesi dei fini - e questa è la lettura benevola - oppure una piccola grande furbizia. Sulla sua motivazione originale non ci sono dubbi, essendo dichiarata dagli stessi promotori della proposta. La norma nasce per salvare dal pagamento di multe anche salate qualche centinaio di cacciatori, in prevalenza trentini, sanzionati perché cacciavano fuori dai loro territori di residenza venatoria (soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano), praticando un'opzione di caccia diversa da quella, chiamata «vagante nelle Alpi», per la quale hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria. suddette multe sono state comminate, malgrado i sanzionati fossero autorizzati a cacciare in trasferta dalle locali autorità venatorie. Sembra una circostanza complicata, ma in realtà non lo è: 157 del 1992 prevede tre forme di caccia (vagante nelle Alpi, da appostamento fisso e generale), da esercitare in forma esclusiva. Se la lingua italiana ha un senso, ciò significa che, se uno pratica la caccia alpina, non può praticare quella da appostamento fisso. Sanzionando queste centinaia di cacciatori sconfinati dal proprio territorio e dalla propria opzione venatoria di riferimento, l'autorità di vigilanza venatoria ha stabilito che l'esclusività dell'opzione di caccia vale anche nel caso in cui si stia cacciando ospitati al di fuori della propria zona zona venatoria, che - lo ricordo - non coincide con la zona di residenza anagrafica: si può essere cittadini trentini e decidere di risiedere dal punto di vista venatorio in Toscana, per esempio; la legge lo consente, e questo è bene ricordarlo e sottolinearlo. Questa è, in sintesi, la premessa da cui nasce questa leggina. Ebbene, tale premessa poteva - forse doveva - dar luogo a una qualche risposta: ma una risposta circoscritta al caso e al problema specifico. Essendo fuori discussione la buona fede dei cacciatori multati, si poteva percorrere una via, amministrativa o legislativa, che, sanando la loro situazione, ribadisse però una volta per tutte ciò che nella legge nazionale, al di là delle acrobazie verbali di qualche collega, è di assoluta chiarezza, se l'italiano ha un senso: ogni cacciatore deve scegliere una e solo una opzione di caccia tra le tre possibili; tale opzione esclusiva vale dovunque egli stia esercitando l'attività venatoria; nessuna legge regionale, o provinciale, come nel caso del Trentino, nessuna Regione o Provincia, per quanto a Statuto speciale, possono derogare da questo criterio, per la semplice ragione che si sta parlando di un tema, la tutela della fauna, che la Costituzione assegna alla potestà esclusiva dello Stato e su cui, dunque, Regioni e Province, anche quelle a Statuto speciale, devono attenersi ai principi fissati nella normativa nazionale. Su tale punto ci sono molte sentenze della Consulta che sono eloquenti da questo punto di vista. Tutto questo non si è fatto. Invece, per condonare duecento o trecento cacciatori, si è scelto di mettere in discussione uno dei principi-cardine della legge n. 157. Prevedere come esclusiva la scelta di una delle tre opzioni di caccia non era e non è né un capriccio del legislatore né un caso: è invece una delle basi di quell'ottima legge; è l'idea che ogni cacciatore debba collegare la propria attività non solo a un determinato territorio, ma anche a una tipologia di esercizio venatorio. È grazie all'affermazione di tale principio che in Italia la caccia non rappresenta una minaccia per la conservazione della fauna selvatica. Colpire questo principio significa favorire il turismo venatorio e la caccia privata a pagamento; significa riaprire lo scontro tra chi vorrebbe semplicemente vietare la caccia e chi la vorrebbe vorrebbe privatizzata e praticata senza regole e senza limiti; significa - aggiungo - rompere la positiva collaborazione che ha visto, in questi ultimi venti anni, la parte più matura del mondo venatorio impegnata fianco a fianco con le associazioni di tutela ambientale per consolidare un modello sostenibile di gestione della fauna selvatica che, lo ricordo (ed è la Costituzione che lo stabilisce), è patrimonio indisponibile della collettività, mentre la caccia - mi dispiace smentire il senatore Carrara - non è un diritto bensì una facoltà che la legge riconosce, entro certi limiti, ad alcuni cittadini. Già all'inizio di questa legislatura la destra provò a fare tutto questo con il disegno di legge che portava la firma del senatore Orsi e che, contro la sensibilità largamente maggioritaria degli italiani, avrebbe aperto la strada a una sorta di caccia «*no-limits*». Quel tentativo fallì per l'opposizione nostra, di

Grazie, qualche reduce o qualche nostalgico, anche presente in quest'Aula, questa norma abbia il senso di riprodurre, seppure in sedicesimo, quella stessa operazione. Anche per questo, oltre che per la vistosissima sproporzione tra i fini che si propone il disegno di legge Divina e i mezzi adottati per raggiungerli, noi voteremo contro.

intervengo molto brevemente. Rifacendomi alle valutazioni ottimamente espresse dal senatore Orsi, nostro Capogruppo in Commissione ambiente, e dal relatore, senatore Molinari, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà su questo disegno di legge, interpretativo di una piccola porzione della legge n 157 del 1992, che rende giustizia a qualcuno che aveva subito una cattiva interpretazione

So che nessuno di noi può evitare di provare un indicibile strazio al pensiero di quella ragazzina di 14 anni che era appena tornata da scuola per andare incontro alla sua morte. Tuttavia, verremmo meno al nostro dovere se esprimessimo per queste vittime un generico cordoglio, se chiamassimo in causa solo il destino e la fatalità, perché questa è anche una tragedia del lavoro, una tragedia delle donne, una tragedia del Sud, una tragedia che deve scuotere le nostre coscienze, aiutarci a compiere meglio il nostro dovere, a meglio tutelare e proteggere la comunità che siamo tutti chiamati a servire. La magistratura naturalmente chiarirà quali responsabilità colpose possano esserci dietro l'accaduto, ma nel frattempo è potente la suggestione che porta ad accostare queste quattro operaie morte sul lavoro a quelle arse nell'incendio della loro fabbrica: anche quella - a New York, un'azienda tessile. Ed è più di una suggestione: è la consapevolezza che la crisi, prima di essere una questione di *spread*, di *rating*, di *default* e di *dumping*,è una questione di lavoro ingrato, di salari compressi e saccheggiati, di tutele allentate e diritti negati. Alle donne, specialmente nel Mezzogiorno, tocca in sorte di essere ultime fra gli ultimi, debolissime fra i deboli. È una tragedia del Sud, dell'assenza e della debolezza dei poteri pubblici. Il crollo di Barletta è l'ultimo, in ordine di tempo, di un rosario di dolore e di lutto che sembra infinito, che si snoda attraverso lo spaventoso eccidio che avvenne nella stessa Barletta 52 anni fa, il crollo di Castellaneta del 1985, l'immane tragedia di viale Giotto (nella mia Foggia) di quasi 12 anni fa, dove perirono 78 persone, per limitarmi solo agli episodi più tragici. È una geografia che, con poche eccezioni, si ferma a Roma, ed è difficile credere ad una fatalità che segue l'andamento dei paralleli. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il cupo fragore di quel crollo, le macerie e i detriti di Barletta rischiano di non riguardare solo quella palazzina, quelle povere persone e quella bella città. In questo momento di dolore e smarrimento è forte il timore che, in esso, si rispecchi il crollo dell'aspirazione di tutti noi ad un Italia più unita e più giusta, alla piena realizzazione del precetto costituzionale che definisce la nostra Repubblica una, indivisibile e fondata sul lavoro. Da donna, da meridionale, da parlamentare, supplico tutti voi, in questo giorno di sofferenza e di lutto, di non risparmiare sforzo alcuno affinché il disegno affidatoci dai nostri maggiori sia compiuto e non rinnegato. Vi ringrazio.

Non possiamo che stringerci attorno alle famiglie di quelle cinque persone, di cui una bambina, ed essere vicino a loro, sperando che in questo momento, di fronte alla tragedia,

perché veniamo presi contemporaneamente da sconforto, da rabbia, da cordoglio e assaliti da una serie di interrogativi. Come mai ancora non riusciamo ad evitare queste tragedie incredibili, che segnano non soltanto le vite disgraziate rimaste seppellite sotto le macerie,

i morti sul lavoro; ci siamo impegnati tutti quanti, abbiamo discusso su un problema serissimo, una situazione drammatica, che però drammaticamente si ripete.

che ripetutamente accadono. Noi siamo costernati e addolorati per quello che è successo, ma questo non basta più. C'è bisogno di un intervento legislativo, economico e finanziario, che ponga fine a questa tragedia.

Signora Presidente, anch'io mi associo al cordoglio espresso dai colleghi per le vittime del grave episodio che si è Ieri, Presidente, nel nostro Paese si sono verificati tre avvenimenti molto gravi, a mio avviso. Il primo è quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Il secondo è l'uscita della FIAT da Confindustria, cosa che testimonia un livello di malessere evidente nel mondo imprenditoriale, soprattutto in quello della grande impresa, in particolare se leggiamo questo episodio insieme al comunicato di Della Valle relativo alla situazione delle imprese italiane. lo scollamento che si è verificato all'interno di Confindustria sia meritevole di attenzione. Ho la sensazione, infatti, che ci sia l'esigenza di offrire alle piccole e medie imprese una sponda di natura politica necessaria

Mi auguro che ci sia qualcuno che si ponga il problema della figura che ha fatto il nostro Paese in questa vicenda. Mi auguro che non ci sia più carcere se non ci sono prove. Mi auguro che non ci sia più carcere per estorcere la verità, una verità di comodo, funzionale ai teoremi che vengono ideati. Mi auguro che non ci sia più carcere

ad indagare sulla base di prove documentate e non di prove estorte attraverso una forzatura della detenzione preventiva, attraverso una forzatura degli strumenti processuali, attraverso una carcerazione ingiusta che determina, purtroppo, fenomeni come quello che tutti abbiamo visto ieri attraverso i teleschermi.

della Presidenza e delle Commissioni parlamentari la gravissima scorrettezza alla divulgazione della famosissima lettera della BCE firmata dai signori Draghi e Trichet con la quale l'Italia è stata commissariata. Riepiloghiamo. Il 5 agosto la Banca centrale europea invia una lettera di vero e proprio commissariamento dell'Italia, della sua politica economica, che ha costretto il Parlamento a varare l'ennesima «manovra lacrime e sangue» da 60 miliardi di euro, dopo le precedenti, per rassicurare i mercati i quali, ciò nonostante, hanno continuato a registrare speculazioni sui titoli di Stato, facendo segnare i titoli del debito pubblico italiani e i *Bund* tedeschi che viaggia tra i 370 e i 430 punti base. Tale speculazione dei mercati, in parte raffreddata dagli interventi di acquisto dei BTP, si traduce in un aumento dei tassi di interesse per rifinanziare i titoli del debito pubblico. ciò ha portato molti parlamentari nelle Commissioni competenti, tra le quali la Commissione finanze e la Commissione bilancio (che ha dovuto lavorare quest'estate), a chiedere conto al Governo di questa famosa lettera. Il Parlamento ha dovuto deliberare al buio, senza conoscere i motivi del commissariamento. Ora, signora Presidente, ritengo che lei si debba cortesemente fare carico della mia richiesta al presidente del Senato, perché non è possibile che, come si faceva tempo fa, con l'agenzia Stefani di un passato regime che ci auguriamo non torni più, i Ministri economici di questo Governo, gli stessi che sono garanti, con lo scudo fiscale, degli evasori fiscali, che hanno fatto un vero e proprio riciclaggio di Stato, neghino la lettera al Parlamento, alle Commissioni parlamentari, alla Presidenza di quest'Aula e passino le veline ai giornali e ai giornalisti amici. Se questa cosa passa sotto silenzio, noi dell'Italia dei Valori la portiamo all'attenzione di quest'Aula, perché riteniamo che sia indecente e scorretto che vengano passate le veline a giornalisti amici, come accadeva in passato, per diffondere per diffondere ad orologeria documenti apparentemente coperti e poi desecretati *ad hoc* per fini di lotte politiche all'interno della maggioranza. La prego, signora Presidente: il Parlamento è una cosa seria, non un orpello a disposizione dei Ministri e del Governo di turno. Quando i parlamentari chiedono nelle apposite Commissioni di conoscere per deliberare, ciò viene loro negato, e poi essi si ritrovano questa lettera pubblicata sul «Corriere della Sera». Ebbene, io ritengo che bisogna ribellarsi a quest'offesa: